a causa del ritardo con cui viene data, perde un po' di valore, avendo il direttore generale Francesco Micheli assunto la decisione di rimettere l'incarico di direttore dell'azienda di trasporto

L'interrogazione richiede chiarimenti sulle procedure che hanno consentito all'azienda di affidare l'incarico di direttore generale ad un soggetto in quiescenza, nello specifico al dottor Francesco Micheli, viste le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplina la fattispecie riguardante il divieto, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT e per le autorità indipendenti (queste sono le tre fattispecie cui la norma si applica), di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza. Segnalo che sul tema il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato apposite circolari (la n. 6 del 2014 e la n. 4 del 2015), che hanno proprio lo scopo di rafforzare e precisare l'ambito di applicazione della norma contenuta nell'articolo 5 citato. Le predette circolari ribadiscono il divieto di conferire incarichi a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza, indipendentemente dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza. circolari si chiede esplicitamente alle amministrazioni di evitare comportamenti elusivi consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza. Per tali soggetti le amministrazioni possono valutare la possibilità di conferire un incarico gratuito, ma su questo tornerò in seguito. La *ratio* della norma risiede nell'esigenza di impedire che le amministrazioni pubbliche continuino ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza, attribuendo loro rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto e impedendo che incarichi di vertice vengano conferiti a dipendenti più giovani, con il rischio che, con il permanere in servizio, vi sia anche una continuità a volte non sempre trasparente. La norma quindi mira ad agevolare sia il ricambio che il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Come altre disposizioni vigenti che già limitavano la possibilità di conferire incarichi a soggetti in quiescenza, contenute nelle leggi di stabilità degli anni precedenti, le citate norme non sono volte ad introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con le esigenze di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa. Le norme infatti consentono di affidare incarichi a titolo gratuito per un anno, proprio con il fine di agevolare il passaggio di consegne e il trasferimento di competenze fra chi esce dall'amministrazione e chi vi subentra. Concludo dicendo che - com'è noto e come ho detto all'inizio - il dottor Francesco Micheli non riveste più la carica di direttore generale e che la competenza del Dipartimento della funzione pubblica e del Governo non ci consente di agire direttamente sulle decisioni che riguardano aziende non inserite nell'elenco ISTAT e di proprietà Ciò non toglie che possano essere attivati altri strumenti per mettere in risalto comportamenti non corretti, quando appunto le situazioni riguardino enti ai quali si applica direttamente la normativa di riferimento e sulle quali il Governo abbia una competenza diretta.

Signora Presidente, qualche tempo fa ha destato sconcerto questa notizia perché, oggettivamente, in tutta la vicenda della Resistenza, chi ha partecipato alla guerra di liberazione stava dalla parte giusta,

detenuti per altri motivi. Il fatto che il responsabile di tale massacro, condannato a morte e poi amnistiato per questa vicenda, Valentino Bortoloso (detto "Teppa"), avesse ricevuto questa medaglia della Resistenza, appunto, ha suscitato grande clamore perché, alla fine, ciò infanga la vera Resistenza. Questo riconoscimento, dato a una persona con quei precedenti, svilisce il sacrificio e l'impegno

Il 25 aprile 2015, in occasione della ricorrenza del 70° anniversario della Guerra di liberazione e della Resistenza, il Ministro della difesa ha inteso conferire ai partigiani, agli ex internati nei *lager* nazisti, nonché ai combattenti inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate ancora in vita una medaglia commemorativa denominata "medaglia della Liberazione". L'iniziativa, fortemente voluta dal Ministro, ha trovato ulteriore supporto in una risoluzione parlamentare, approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati volta a conferire un attestato ai partigiani, ai combattenti, ai patrioti, ai reduci e ai militari che hanno contribuito alla lotta di liberazione. La stessa iniziativa ha riscosso amplissimi consensi su tutto il territorio nazionale e ha registrato una grande partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, a quelle che si sono rivelate vere e proprie feste popolari, contribuendo così a mantenere viva la memoria delle vicende fondanti la nostra Repubblica e a trasmetterne il valore alle generazioni future. Ad oggi, a fronte di tali manifestazioni, nel corso delle quali sono state consegnate circa 6.000 medaglie, il caso evidenziato dal senatore interrogante risulta essere l'unico con profili di criticità. Al riguardo, il 16 giugno scorso si è svolta presso la prefettura di Vicenza la cerimonia di consegna della medaglia della liberazione a 83 partigiani segnalati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dall'Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC), dalla Federazione italiana volontari della libertà dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dall'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla Guerra di liberazione (ANRP) e dall'Associazione nazionale combattenti della Guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate Queste associazioni si sono fatte carico di raccogliere tutte le istanze, verificarne e certificare il possesso dei requisiti degli istanti ed inviarle al Ministero della difesa. Tra gli insigniti era presente anche il signor Valentino Bortoloso. A seguito di approfondimenti condotti dalla Difesa su richiesta delle autorità locali, è stato appurato che l'interessato fu coinvolto in un grave evento delittuoso, richiamato testé dall'interpellante, occorso presso le carceri della città di Schio tra il 6 e il 7 luglio 1945, a seguito del quale subì una condanna in forma definitiva. Per tale ragione, il Ministro della difesa ha deciso di procedere alla revoca della medaglia della liberazione attribuita al Bortoloso e alla conseguente cancellazione del nominativo dall'Albo dei premiati, notificando tale decisione al prefetto di Vicenza ed all'ANPI già in data 5 agosto 2016.

a costo zero, un'idea da coltivare. per quanto concerne le premesse che motivano l'atto di sindacato ispettivo, occorre preliminarmente osservare che, con decreto dirigenziale n. 10 del 5 gennaio 2012, l'interessato veniva escluso dalla procedura concorsuale e dalla relativa graduatoria di merito per difetto delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo del 2001. La legittimità del provvedimento veniva sancita con sentenza n. 5628 del 2012 del TAR del Lazio, poi divenuta definitiva per omessa impugnazione. Pertanto, tra l'interessato e l'amministrazione della difesa non si costituiva alcun rapporto di servizio, suscettibile di reintegro per effetto della sentenza resa dal giudice per le indagini Nel merito della richiesta del provvedimento di reintegro, pur comprendendo l'auspicio dell'onorevole interrogante, esso non è adottabile nel caso in esame. L'amministrazione, allora come oggi, è priva di ogni potere discrezionale nella gestione delle procedure concorsuali e deve invece conformare il proprio operato ai dettato legislativo in virtù del quale, per accedere alla procedure concorsuali e per instaurare un valido rapporto di servizio, è necessario che il concorrente possegga e mantenga continuamente, sino all'immissione in ruolo, i requisiti previsti dal legislatore. Il possesso in via continuativa dei requisiti per costituire il rapporto di servizio, si configura come un principio inderogabile e generale che informa l'intero ordinamento. Di fatto, anche per la costituzione di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione è necessario che il contraente privato abbia e mantenga i requisiti di moralità previsti dal legislatore, non solo durante le fasi della procedura e nella stipulazione del contratto, ma anche sino alla fine dell'esecuzione del rapporto. In relazione ai soggetti coinvolti, trattandosi non di un reintegro in una posizione già posseduta, ma di una immissione in ruolo per il quale il concorrente aveva perso i requisiti di partecipazione, il provvedimento andrebbe altresì ad incidere sul contingente inserito in servizio permanente. Pertanto, il provvedimento richiesto sarebbe affetto da un ulteriore profilo di illegittimità andando a incidere, da allora, sulla graduatoria: andrebbe infatti a ledere le legittime posizioni dei dipendenti già immessi in ruolo e a violare interessi di rango superiore, quali la *par condicio* dei partecipanti al concorso, la stabilità dei ruoli e l'interesse della stessa amministrazione. Neppure l'elemento di novità costituito dalla sentenza del giudice per le indagini preliminari di Nocera Inferiore, passata in giudicato, è in grado di incidere sull'azione amministrativa, in difetto dell'omesso appello al Consiglio di Stato avverso la citata decisione del TAR del Lazio. In relazione a quanto finora esposto, l'amministrazione della difesa appare al momento impossibilitata ad adottare un provvedimento di revoca dell'atto di esclusione a suo tempo adottato. I profili esposti dall'onorevole senatore rendono comunque opportuno esaminare eventuali ulteriori prospettazioni anche per valutazioni più complessive di tali fattispecie compatibili con l'ordinamento militare.

è molto tecnica ed arida e, per alcuni versi, posso dire anche superficiale. Va detto, in maniera secondo me abbastanza forte in questa Assemblea, che la Costituzione e le leggi

e forestali*. Signora Presidente, è esattamente così, come ha appena detto. Signora Presidente, onorevoli senatori, faccio anzitutto presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non svolge attività di vigilanza e controllo sui consorzi di bonifica, funzioni queste espletate dalle Regioni e dalle Province autonome, che li disciplinano con specifiche normative. Ciò posto, preciso che, in base alle informazioni assunte dal Consorzio di Piacenza, l'immobile in questione è di proprietà demaniale ed è stato ad esso affidato per l'esercizio delle pertinenti attività istituzionali. Si tratta, in particolare, di uno stabile preposto al ricovero di materiali, pezzi di ricambio, attrezzature e mezzi necessari al quotidiano svolgimento delle attività di bonifica svolte nell'area Arda-Basso-Piacentino. In tale contesto, il bene viene altresì utilizzato come alloggio di servizio del personale che esercita funzione di custodia e vigilanza del materiale e delle attrezzature ivi depositate. Come precisato dal Consorzio in parola, tale ultimo impiego, oltre ad essere conforme ai propri fini istituzionali, è espressamente contemplato quale forma di retribuzione in natura, dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti dei consorzi di bonifica. Per quanto sopra, il comitato amministrativo competente ha deciso di destinare il bene in questione, anche per il 2016, ad alloggio di servizio del proprio dipendente, individuando un canone forfettario a parziale copertura delle spese (invero esigue) sostenute dal Consorzio per il mantenimento in uso dell'immobile.

e ripresa in diversi articoli di stampa, relativa alla mancata esecuzione di provvedimenti definitivi per l'inadeguatezza delle dotazioni di personale amministrativo registrata nel distretto. Il Ministro della giustizia ha avviato, nell'immediatezza della pubblicazione degli articoli di stampa citati, mirati approfondimenti sui ritardi dell'ufficio esecuzione penale presso la corte d'appello di Napoli, per mezzo delle competenti articolazioni. L'ispettorato generale ha quindi riferito, in una preliminare informativa, che una situazione di criticità era già stata rilevata nel corso dell'ispezione ordinaria eseguita nel 2013. In particolare, i fascicoli in attesa di adempimenti a cura della cancelleria risultavano essere 9.878, di cui 4.370 sentenze, 3.647 procedimenti da restituire al giudice di primo grado, 1.860 restituiti dalla Corte di cassazione e in attesa di essere ritrasmessi al giudice di primo grado e 330 da trasmettere alla Corte di cassazione, essendo stato presentato il relativo ricorso. Analoghi ritardi erano stati rilevati in merito al recupero di spese processuali e pene pecuniarie. Era anche emerso - quanto al ritardo nella compilazione dell'estratto esecutivo per i condannati a piede libero - che, nei casi di condanna a pene severe, la cancelleria aveva provveduto di regola con sollecitudine e, tuttavia, a causa dell'elevato numero di fascicoli, vi era il rischio che sentenze di condanna restassero ineseguite per un tempo eccessivo. L'ispezione, dunque, evidenziò l'esigenza di una redistribuzione del personale tra i vari servizi, in modo da impegnare unità aggiuntive nei settori in sofferenza, nonché di provvedere a un *turnover* delle posizioni lavorative che possono generare *stress*, riducendo la produttività. Tra l'altro, Tra l'altro, analoghe criticità erano state rilevate dall'ispettorato presso altri uffici giudiziari similari, anche di grandi dimensioni, e anche in tali casi specifiche e dettagliate prescrizioni erano state impartite per la normalizzazione dei servizi. Anche per Napoli, pertanto, all'esito dell'ispezione del 2013, fu formulato un preciso invito al capo dell'ufficio ad adottare formali direttive di *governance* necessarie per il superamento dei ritardi, anche attraverso la rivisitazione dei modelli di lavoro e la razionalizzazione distributiva delle risorse umane, oltre che alla verifica dei risultati da conseguire attraverso quelle misure. Sono, quindi, del giugno di quest'anno le dichiarazioni del presidente della corte d'appello di Napoli, secondo le quali sarebbero prive di esecuzione 50.000 sentenze, di cui 30.000 di condanna, e, tra queste ultime, 12.000 sentenze di condanna alla pena della reclusione, recando il residuo condanne a pena di altro genere. Come sopra rilevato, il Ministero ha disposto immediati accertamenti in ordine al volume delle sentenze ineseguite e all'adozione di efficaci modelli gestionali. All'esito di preliminari interlocuzioni, il capo dell'ispettorato e il capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria lo scorso 8 settembre hanno svolto una visita mirata presso gli uffici della corte d'appello di Napoli, a conclusione della quale è stato richiesto al presidente della corte un piano straordinario di intervento urgente, alla cui esecuzione gli uffici ministeriali hanno assicurato ampio sostegno. Peraltro, occorre rilevare che i presidenti delle corti d'appello, per fronteggiare situazioni di criticità, dispongono, nell'esercizio dei loro poteri di sorveglianza, delle misure dei comandi e delle applicazioni di personale del distretto. L'effettiva attuazione del piano straordinario, da adottarsi con l'urgenza del caso, sarà perciò monitorata con estrema attenzione dal Ministero, anche al fine dell'esercizio delle sue prerogative. In generale, anche in questa sede va ribadito che il Ministero ha posto al centro della sua attenzione il personale amministrativo presso gli uffici giudiziari italiani, al fine di assicurare agli stessi tale fondamentale supporto. Il lavoro di questi anni ha consentito di raggiungere importanti risultati e di tracciare nuovi percorsi, nel cui solco occorre continuare ad indirizzare l'azione amministrativa del Ministero. Si ricordano in particolare in tale contesto le misure straordinarie per il reclutamento di nuove risorse, con il bando per mobilità volontaria per 1.031 posti pubblicato il 18 febbraio 2015, e le procedure di mobilità obbligatoria promosse in attuazione delle leggi di stabilità per per il 2015 e per il 2016; l'avvio delle procedure di riqualificazione autorizzate dall'articolo 21-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2015, che consente il passaggio di area alle due fondamentali qualifiche di cancellieri e ufficiali per nel novembre 2015, dell'accordo sul Fondo unico di amministrazione, con il quale sono stati finalmente redistribuiti 90.496.445 di euro relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, destinati a tutto il personale del Ministero, e nel quale proprio per il personale dell'amministrazione giudiziaria è stato delineato, per la prima volta, un sistema graduale di introduzione di meccanismi premiali. A tali obiettivi si sono aggiunte le fondamentali misure introdotte dal decreto-legge n. 117 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 161 dell'agosto 2016, con il quale si è conseguito il significativo risultato dell'ingresso di nuove risorse negli uffici giudiziari, mediante procedure di assunzione, che aprirà al processo di ringiovanimento di passaggio di competenze professionali nell'amministrazione giudiziaria da molti anni atteso. Si tratta di un programma articolato di assunzioni, con l'immediato reclutamento a tempo indeterminato di mille nuove unità di personale amministrativo non dirigenziale, cui potranno aggiungersi ulteriori, ancor più significative risorse una volta completate le procedure di mobilità obbligatoria. Con il decreto citato si raggiunge non soltanto il fondamentale obiettivo dell'avvio di nuove assunzioni, dopo anni di sostanziale stagnazione delle fonti di reclutamento concorsuale, La norma prevede, infatti, la possibilità di introdurre nuovi profili, anche tecnici, e di rimodulare e rivedere i profili professionali e i relativi contingenti esistenti, prioritariamente per far fronte alle nuove e accresciute competenze dell'amministrazione collegate al trasferimento delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari e al rinnovato impulso dei processi di digitalizzazione avanzata. L'autorizzazione alla revisione delle dotazioni organiche delle singole aree con un procedimento semplificato permette, poi, di accompagnare le procedure di reclutamento per mobilità e quelle di riqualificazione in modo coordinato e coerente con l'apporto di nuove risorse che dalle assunzioni scaturirà. Il Ministro ha tracciato le linee di intervento per il personale dell'amministrazione giudiziaria con la propria direttiva dell'8 settembre scorso, al fine di assicurare al nuovo personale la più idonea e adeguata formazione, valorizzando le competenze già diffuse nei vari uffici sul territorio e facendo ricorso a più innovativi e agili strumenti di formazione. Nel quadro complessivamente tracciato in una situazione generale di scarsità di risorse umane, il Ministero ha prestato particolare attenzione agli uffici del distretto della corte d'appello di Napoli, proprio in considerazione della complessiva situazione riscontrata. Il Ministero ha provveduto, difatti, ad assegnare sin dal 2014 agli uffici 24 funzionari, su un totale nazionale di 138 disponibilità, a seguito di un accordo di condivisione delle graduatorie relative a concorsi banditi dall'Istituto per il commercio con l'estero e dal Ministero dell'interno. Anche in seguito alle procedure di mobilità volontaria, sono stati pubblicati 116 posti, di cui 28 sono stati coperti. Ulteriori posti sono stati resi disponibili attraverso le procedure di mobilità obbligatoria di mobilità obbligatoria di cui alla ricordata legge di stabilità per il 2015, attraverso lo speciale portale gestito dal dipartimento della funzione pubblica. Infatti, a fronte di un totale complessivo di 104 posti offerti nel distretto di Napoli, vi sono state 54 opzioni da parte di personale che deve essere ricollocato. Al momento attuale, al distretto della corte d'appello di Napoli risultano assegnate dotazioni in pianta organica pari a complessive 4.241 unità, di cui 3.450 risorse presenti.

Occorre con chiarezza evidenziare - diversamente da quanto rappresentato nell'interrogazione - che l'attuale assetto delle piante organiche del personale amministrativo è stato determinato, con i decreti ministeriali del 25 aprile 2013 e del 19 maggio 2015, tenendo conto dei carichi di lavoro rilevati in epoca immediatamente anteriore. Pertanto, la pianificazione dei fabbisogni di personale amministrativo è stata elaborata a conclusione del processo di revisione della geografia giudiziaria, avviato nel 2012, considerando opportunamente i nuovi assetti, in termini di risorse, conseguenti all'accorpamento degli uffici. La situazione degli uffici, sia quanto al personale di magistratura che amministrativo, è stata oggetto di un costante monitoraggio e, all'esito della disponibilità dei dati statistici consolidati riferiti agli anni successivi all'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria e di una approfondita analisi degli elementi degli elementi idonei a rappresentare le effettive esigenze operative dei presidi giudiziari, è stata elaborata dagli uffici del Dicastero una proposta di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado, ora all'esame del cui seguirà la coerente revisione dei fabbisogni di personale amministrativo. Nella elaborazione delle nuove piante organiche del personale amministrativo si dovrà tener conto della semplificazione strutturale delineata nel nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Infine, la maggiore efficienza operativa, realizzata anche attraverso l'unificazione della gestione dei beni e dei servizi serventi l'amministrazione centrale e gli uffici periferici, consentirà di corrispondere con maggiore tempestività alle esigenze degli uffici giudiziari, sostenendo il processo di rinnovamento dei relativi assetti organizzativi e la crescente informatizzazione di tutti i servizi inerenti l'amministrazione della giustizia. Al fine Al fine di dare effettività a tutte le misure organizzative già adottate e di prossima adozione, saranno quindi individuati, nell'ambito della nuova dotazione complessiva, i contingenti delle singole professionalità, anche di nuova istituzione, che saranno successivamente ripartiti tra gli uffici giudiziari e le strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione giudiziaria.

linguaggio burocratico, rinvia ad eventi futuri e abbastanza incerti e non risponde nello specifico, perché non dettaglia

Qui c'è un problema, un problema grosso: si tratta di migliaia di sentenze non eseguite, di gente che non va in carcere e noi ancora non sappiamo di chi sia la responsabilità di tutto questo e da che cosa sia stato causato.

Signora Presidente, mi riferisco all'interrogazione con la quale la senatrice Puppato chiede al Ministero notizie in merito al monastero benedettino dell'Abbazia di Sant'Eustachio sita a Nervesa della Battaglia, in Provincia di Treviso ed in particolare circa l'affidamento dei lavori da parte del Comune di Nervesa della Battaglia, nelle more dell'*iter* di accertamento sulla procedura ad evidenza pubblica concernente la concessione della progettazione esecutiva, del restauro e del recupero architettonico e strutturale dell'abbazia, ancora in corso, da parte di ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui sono subordinati la definitiva stipula contrattuale e la conseguente consegna ed avvio dei lavori. Occorre premettere che l'immobile è stato dichiarato di interesse culturale, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 10, commi 1 e 12, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), con provvedimento del 13 marzo 2014. L'immobile appartiene al Comune di Nervesa della Battaglia, in Provincia di Treviso che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 55 del codice (che disciplina l'alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali), ha inoltrato alla competente Soprintendenza, nel maggio del 2016, istanza di autorizzazione alla concessione in uso, ai sensi del secondo comma dell'articolo 57-*bis* dello stesso codice, che prevede appunto la possibilità che i beni del demanio culturale possano essere locati o concessi in uso. L'autorizzazione richiesta dal Comune è stata oggetto di valutazione collegiale in data 9 giugno 2016 della Commissione regionale per il patrimonio culturale. Il Collegio ha esaminato il caso sulla scorta del parere istruttorio espresso nel merito dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, ed ha formulato il provvedimento di autorizzazione al trasferimento del bene mediante concessione in uso, ai sensi del comma 3 del sopra citato articolo 55 del codice, dettando le seguenti prescrizioni e condizioni. luogo, alla voce «prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate», è stabilito che la conservazione del bene sarà assicurata mediante adeguati provvedimenti restaurativi, con particolare riferimento all'architettura del monumento e alle aree scoperte di pertinenza. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza competente ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere storico o artistico dell'immobile, escludendo ogni pregiudizio alla sua conservazione. Alla «condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso», il provvedimento dispone che le modalità di fruizione pubblica saranno quelle consentite dalle previste destinazioni d'uso culturali, espositive e didattiche, coincidenti in particolare con la conservazione e la fruizione del monumento, e alle sue condizioni di decoro. Infine, alla voce «congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta», si considerano congrui gli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta di autorizzazione alla concessione in uso ed il termine di cinque anni decorrenti dalla data di concessione in uso per il loro conseguimento. Il provvedimento è stato emanato nell'ambito della competenza autorizzatoria di cui agli articoli 55 e seguenti del codice e, conseguentemente, non entra nel merito del termine di ottanta anni di durata della concessione, che è argomento che esula dalla materia della tutela, ancorché connesso ai tempi di realizzazione e dell'impegno finanziario che gli obiettivi di valorizzazione richiedono. La materia, infatti, è più propriamente riferita alla sfera della libertà di mercato e della difesa della libera concorrenza. Infatti, la questione è stata sottoposta all'Autorità nazionale anticorruzione che, nella recente deliberazione in data 5 luglio 2016 (deliberazione che, in effetti, la senatrice interrogante non poteva conoscere, perché la data della deliberazione dell'ANAC coincide con quella di presentazione dell'interrogazione), ha ritenuto di non ravvisare margini per un proprio intervento. Concludo precisando che, in ogni caso, l'esecuzione del progetto allegato all'istanza di concessione rimane sottoposta alla competenza della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *b)*, del codice; in base al quale le Soprintendenze «autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni cultural», ed esercitano altresì tutte le facoltà, attribuite loro dalla parte seconda del codice stesso, di vigilanza, ispezione, protezione e conservazione del bene culturale.

Faccio presente che, naturalmente, vigileremo, perché stiamo parlando di una concessione che in termini temporali è molto più assimilabile a un diritto di superficie (che sappiamo essere

si proceda con tanta celerità, senza prima attendere, come sarebbe stato obbligatorio e più che opportuno, i pareri degli enti competenti. Vigileremo comunque perché l'utilizzo del bene pubblico mantenga